Comunico che in data 21 dicembre 2023 è stato presentato il seguente disegno di legge: *dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dal Ministro della difesa* «Conversione in legge del decreto-legge 21 dicembre 2023, n. 200, recante disposizioni urgenti per la proroga dell'autorizzazione alla cessioni di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina»

Comunico che è pervenuto ed è in distribuzione il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sull'emendamento 1.9000, interamente sostitutivo degli articoli della prima sezione del disegno di legge. Come stabilito dalla Conferenza dei Capigruppo, si passerà direttamente alle dichiarazioni di voto sulla fiducia. Avverto che è in corso la trasmissione diretta televisiva. Invito pertanto i colleghi che interverranno in dichiarazione di voto

dovuto essere una manovra impeccabile, non solo dal punto di vista dei contenuti ma anche della procedura. In realtà questo assunto è crollato rapidamente. La manovra inemendabile è stata ripetutamente emendata, i tempi si sono allungati, i malumori interni alla maggioranza sono abbastanza

C'è stato però nel metodo e nel contenuto un risultato significativo che non è ascrivibile alla maggioranza, ma a tutti i Gruppi di opposizione. Mi riferisco alla scelta alla scelta di non disperdere le risorse in mille rivoli, ma di destinare 40 milioni di euro ad un fondo contro la violenza sulle donne. È una scelta importante, una scelta doverosa, una scelta per la quale ringrazio tutti i componenti della Commissione bilancio, in particolare il collega Tino Magni del Gruppo AVS, Marco Lombardo e tutti i componenti della Commissione che hanno fatto un ottimo lavoro. Destinare risorse per potenziare i centri antiviolenza e le case rifugio, per fare in modo che ci sia formazione per gli operatori e per il reddito di libertà è una battaglia che da sempre, come Azione, con Mara Carfagna ed Elena Bonetti, portiamo avanti e di cui siamo profondamente orgogliose.

tale crescita dipendono la qualità dei salari e il benessere di famiglie e imprese. C'è un grande assente in questa manovra di bilancio: il diritto alla salute. Non c'è nessuna attenzione al tema della sanità. Il Ministro ha rivendicato maggiori risorse, ma quelle stanziate non sono sufficienti nemmeno per far fronte al caro energia, all'aumento del costo delle materie prime e dell'inflazione. Si potevano fare tante cose per la sanità, per garantire agli italiani il diritto alla salute, dopo la bocciatura del MES sanitario, ma si è preferito non fare praticamente nulla. Resta inevaso il tema delle liste d'attesa, nessuna risoluzione per il tema dei pronto soccorso, gli italiani continuano a spendere di tasca propria 40 miliardi per potersi curare. Si aspetta anche un anno per la mammografia piuttosto che per un esame istologico e tutto questo è davvero inaccettabile. Con Giusy Versace avevamo proposto di rifinanziare un fondo per per gli ausili e per le protesi, ma anche di questo fondo non vi è alcuna traccia. Per quanto riguarda la famiglia non abbiamo difficoltà a riconoscere che la maggioranza, il Governo ci ha messo delle risorse, ma contestiamo il come vengono investite, perché la platea delle beneficiarie è veramente limitata a coloro che hanno un lavoro a tempo indeterminato. Vi siete completamente dimenticati delle donne lavoratrici autonome, delle partite IVA o di chi, all'interno della pubblica amministrazione, ha ha un lavoro precario. E poi, francamente, la scelta di raddoppiare l'IVA sui prodotti per l'infanzia fa a pugni con le promesse, gli *slogan* e i *social*.

Anche sul tema del rientro dei cervelli, la rimodulazione a fine anno degli incentivi fiscali è un modo per rendere ancora più rigido il sistema italiano.

e profonda di quelli che sono i nostri indirizzi, di quella che è la nostra voglia di incidere fortemente sulla società. Lo facciamo con dei provvedimenti, pur nelle ristrettezze di quella che è una manovra che avremmo voluto fare in maniera completamente diversa, con più fondi a disposizione. Anche le scelte del passato ci hanno costretto a doverci "accontentare" di quello che c'è a disposizione in questo momento. Lo facciamo in maniera netta e decisa, decisa, indirizzando la nostra azione sul sostegno alle fasce più deboli del nostro Paese perché pensiamo che sia fondamentale sostenere ed aumentare la capacità di acquisto delle famiglie,

favorendo anche il fatto che si possa aumentare quella che è la spesa e quindi un ritorno immediato per lo Stato. Sono provvedimenti che hanno un'unica grande direzione. Tutti i parametri economici ci dicono che siamo sulla giusta strada e quindi continueremo in questa direzione, consapevoli del fatto che questa è solo la nostra prima manovra finanziaria, ma che noi abbiamo un compito ben preciso da portare a termine nel quinquennio. Siamo un Governo politico che ha una direzione, che ha una visione e che ha cinque anni a disposizione per intervenire in maniera pesante sulla nostra società, per farla crescere e per arricchirla. Partivamo - come dicevo - dal taglio dal taglio del cuneo contributivo di 7 punti percentuali per tutti i redditi fino a 35.000 euro, che generano comunque un ritorno sulle buste paga con una media superiore ai 100 euro a lavoratore.

portare una decontribuzione fino al 130 per cento per le nuove assunzioni tutte a tempo indeterminato,

perché noi distinguiamo quelli che possono lavorare da quelli che non possono lavorare. Fermo rimane il nostro sostegno alle persone in difficoltà che non possono lavorare, ma attraverso l'eliminazione del reddito di cittadinanza abbiamo incentivato l'occupazione, portando portando le detrazioni al 130 per cento per quelle aziende che investono sui lavoratori, sulla forza lavoro, sulla crescita della forza lavoro e sulla formazione. Sono tutti provvedimenti che portano concreti vantaggi per il lavoro in Italia, perché non esiste non esiste *welfare* che tenga se non c'è un'economia reale che lo sostiene, non esiste una possibilità di sostegno da parte dello Stato se effettivamente non esiste un'economia reale che fa crescere questo Paese, che dà la possibilità di un aumento del PIL, che dà la possibilità di togliere di togliere dall'afasia totale quei ragazzi che non riescono a trovare un posto di lavoro e che solo attraverso l'occupazione possono avere un'identità all'interno di questa nostra società. Un aspetto fondamentale e importante sul quale abbiamo puntato, che faceva parte del nostro programma, è il sostegno alla natalità. Questa è una priorità che avevamo annunciato da tempo

decontribuzione per le mamme lavoratrici e l'aumento del contributo per gli asili nido, perché ogni mamma deve avere la possibilità di scegliere se lavorare o meno e non essere costretta a smettere di lavorare perché non ha la possibilità di poterlo fare.

per le famiglie monogenitoriali con più figli a carico, dando un sostegno importante sempre al concetto di famiglia. Penso che siano tutti provvedimenti di fondamentale importanza, ma non ci sono solamente questi.

lo stanziamento di 5 miliardi di euro per il rinnovo dei contratti di tutti i dipendenti che avevano contratti bloccati da tantissimo tempo.

di discussione generale, pertanto ora mi concentrerò su alcune specifiche questioni che come autonomie abbiamo provato ad affrontare. Il nostro Gruppo ha convintamente sostenuto la proposta di destinare interamente la quota riservata alle opposizioni alla lotta contro la violenza sulle donne. Al di là della cifra, che è comunque significativa, è importante il messaggio alla base, come avevamo già denunciato nell'ultimo intervento normativo, quello che puntava a colmare le lacune del codice rosso, estendendo una serie di misure di prevenzione e protezione; una legge sicuramente ottima, ma fatta a invarianza finanziaria e quindi senza la possibilità di acquistare nuovi braccialetti elettronici o di immettere nuove risorse nel sistema giudiziario. Contro la violenza, infatti, noi possiamo scrivere le leggi migliori del mondo, ma se poi non finanziamo la formazione degli operatori sociosanitari, la costruzione di nuove case rifugio, se non accompagniamo concretamente le donne nella fuoriuscita dai contesti di violenza, le leggi restano lettera morta. L'altro aspetto che mi preme evidenziare, signor Presidente, riguarda il nostro emendamento, assorbito da una proposta dei relatori, che destina 500.000 euro a Trento capitale europea del volontariato 2024. A poche settimane dalla cerimonia di inaugurazione, con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il Comune dispone finalmente delle risorse per questo importante evento, che non ha una dimensione locale ma internazionale e rappresenta un importante riconoscimento per le tante donne, i tanti uomini, i tanti ragazzi e anche i tanti anziani che sono quotidianamente impegnati nelle attività di volontariato, che sono in molti casi una parte importante per il *welfare* del terzo settore. A questo si aggiunge un ordine del giorno che impegna il Governo a stanziare ulteriori risorse per eventuali opere di riqualificazione del patrimonio pubblico collegato alle manifestazioni. Ci tengo, in proposito, a ringraziare tutti i colleghi della Commissione e i relatori che hanno capito l'importanza e l'urgenza del finanziamento, a partire dalla relatrice, la collega Testor, con cui abbiamo fatto un bel gioco di squadra nell'interesse dell'Italia per avere un evento che vedrà al centro della scena europea il terzo settore italiano e del Trentino. Questi interventi sono un buon esempio del ruolo del Parlamento e dei parlamentari sulla legge di bilancio. Quello che fa il Parlamento non è, come crede qualcuno o come qualcuno o come qualcuno cerca di far credere, un assalto alla diligenza, ma il farsi carico di istanze concrete che spaziano dall'interpretazione autentica delle norme al superamento di iniquità che si sono sedimentate nei meccanismi fiscali. Per questo continuo a reputare assurdo l'invito del Governo a non presentare emendamenti: questo ha privato non solo i colleghi della maggioranza, ma anche i territori e le categorie che li hanno eletti della possibilità di vedere rappresentate le loro istanze. Tutto questo ha reso più complicato il lavoro, ma soprattutto ha privato il Senato della possibilità di affrontare temi meritevoli almeno di una discussione. Possiamo comunque dire che l'intera Commissione bilancio ha lavorato con impegno e serietà, a partire dal suo Presidente fino a tutti i suoi componenti. Spero che questo modo di fare la manovra di bilancio non diventi un precedente, perché sarebbe molto grave. Il Gruppo per le Autonomie manterrà, come sempre, un atteggiamento fermo e rigoroso, ma costruttivo nell'interesse del Paese. Signor Presidente, Ministro dell'economia, membri del Governo, onorevoli colleghi, ci sono tre motivi per cui voteremo convintamente contro il vostro disegno di legge di bilancio. Il primo è che è una manovra di bilancio che si basa su un assunto falso; se fosse un'azienda privata sarebbe falso in bilancio. Il secondo è che è una manovra sbagliata nel metodo e nel merito.

Il ministro Giorgetti ha firmato il Patto di stabilità, nel quale c'è scritto che dobbiamo avere una curva di rientro della traiettoria debito-PIL dell'uno La legge di bilancio prevede per i prossimi tre anni una curva di rientro dello 0,1 per cento. La differenza sono 17-18 miliardi di euro all'anno. Per quest'anno, nei numeri che votate oggi - segnatevelo - mancano 18 miliardi. per chi ci segue da casa: tranquilli, la manovra correttiva la faranno dopo le europee, ma quello che è certo è che approvate una legge di bilancio che non sta in piedi. E non date la colpa all'Europa, perché che il Patto di stabilità fosse da rivedere lo sapevamo tutti, lo sapevate voi. La Presidente del Consiglio ha chiuso la sua campagna elettorale dicendo: sul bilancio in Europa la pacchia è finita. Dalla pacchia siete passati al pacchetto. Avete proposto il pacchetto. Il pacchetto non vi ha funzionato e vi hanno dato il pacco e a quel punto il MES è la ripicca. Pacchia, pacchetto, pacco, ripicca: la politica diplomatica e di bilancio del Governo Meloni spiegata in due parole. E mentre da Atreju la Presidente del Consiglio esprimeva le proprie valutazioni sulla rilevante questione del pandoro *gate*, evidentemente immaginando che la sua *leadership* fosse messa in discussione da un'altra *influencer*, il Ministro dell'economia tedesco e il Ministro dell'economia francese chiudevano il pacco-pacchetto-pacchia-ripicca. Il secondo punto è che è un disegno di legge di bilancio sbagliato nel metodo, prima che nel merito. Mi permetta, signor Presidente, per suo tramite, di rivolgermi ai colleghi della maggioranza. Devo essere sincero: ci sono, all'interno delle compagini della maggioranza, personalità

provo emozione perché sappiamo cosa vuol dire stare sul pezzo con i cittadini. Vi sono imprenditori che, da zero, hanno fondato aziende. Poi le hanno vendute, hanno creato posti di lavoro, le hanno fatte ripartire. C'era tanta gente che poteva dare un contributo a questa manovra di bilancio. Voi avete accettato il *Diktat* del Presidente del Consiglio di non presentare emendamenti, con una procedura che è scandalosa. Amici della maggioranza, il vostro Presidente del Consiglio, quando era *leader* dell'opposizione, urlava contro il Governo, dicendo che la democrazia parlamentare era a rischio perché non c'era il tempo per discutere. Mai, però, un Presidente del Consiglio si era permesso di dire: non presentate emendamenti. Questo è il superamento del principio di separazione dei poteri tra legislativo ed Esecutivo. Accettando, avete fatto male al Paese, perché molti di voi sono decisamente più competenti dei tecnici della Ragioneria generale Molti di voi, sulle infrastrutture, sui cantieri, sullo stato di avanzamento dei lavori, su Industria 4.0 potevano dare dei contributi importanti. Avete invece accettato di fare un passo indietro. L'emendamento chi l'ha presentato? L'ha presentato il Governo,

di altri milioni di euro i propri uffici di diretta collaborazione. Ma cosa se ne fa di milioni di euro chi lavora alla diretta collaborazione di Lollobrigida? Gli controlla l'orario dei treni? Cosa può fare la diretta collaborazione a Lollobrigida?

sui pannolini, sugli assorbenti, sui passeggini. Questo è il vostro modo di difendere la famiglia: pensa se non la difendevate! Sulla patria avete detto: bloccheremo i nuovi ingressi. Avete raddoppiato gli sbarchi, ma avete bloccato il rimpatrio dei cervelli.

speravo di poterlo fare senza una previsione normativa. Indipendentemente da questo, se proprio volete suscitare la domanda di senso e di significato di un giovane: perché nel 2023 nel 2023 e nel 2024, nelle vostre due leggi di bilancio, in totale per la 18app, che porta un ragazzo a entrare in un museo, in un teatro, in una libreria, a farsi delle domande di senso profondo della vita, siete passati dai nostri 460 milioni su due anni ai vostri 190 milioni di euro? Il vostro sguardo sulla realtà è uno sguardo che cozza con i numeri e non avete elementi per rispondere nel merito. C'è poi il terzo e ultimo punto, che è quello politico e ho bisogno del MES per parlarne. Il Meccanismo europeo di stabilità era la conclusione per voi dell'accordo sul Patto di stabilità. Vi è saltato Vi è saltato ed essendovi saltato si è prodotta una divisione. Ora io non ho niente da dire né a Fratelli d'Italia né alla Lega. È vero che il MES nasce con il Governo Berlusconi, che la Lega sosteneva e di cui la Meloni faceva parte. Però è anche vero che negli ultimi anni Fratelli d'Italia e la Lega avevano sempre detto che non avrebbero votato il MES. Ho da dire due cose e ne ho da dire anche al MoVimento 5 Stelle. Giuseppe Conte passa dall'essere quello che firma quando è al Governo a quello che attacca quando è all'opposizione: non c'è niente di nuovo nell'atteggiamento del presidente Conte. Lo ha fatto con il decreto Salvini sugli immigrati. Lo può ben fare sul MES. Ho da dire due cose, una a Forza Italia e una al PD. signor Presidente, che il voto sul MES di astensione tradisce una storia, la vostra storia, che nasce a livello europeo nel momento in cui Berlusconi, facendo un'operazione straordinaria, d'accordo con Helmut Kohl, José Maria Aznar, (giganti rispetto ai politici di oggi), e con l'aiuto del Segretario del PPE, Alejandro Agag, decide di portare Forza Italia nel PPE, buttando fuori peraltro il PP di allora. Quella scelta di Silvio Berlusconi è stata una scelta straordinariamente lungimirante, perché ancora Forza Italia all'europeismo. Io poi non l'ho mai votato Berlusconi, ma gli ho sempre riconosciuto questa capacità intelligente di interpretare l'europeismo. Con il voto di astensione sul MES - e capisco l'imbarazzo del collega Gasparri - state tradendo l'eredità politica e culturale di Silvio Berlusconi e dovreste vergognarvi di fronte a quello che è il Partito popolare europeo! PRESIDENTE. Per favore, lasciate intervenire il senatore Renzi. RENZI *(IV-C-RE)*. Chiedo soltanto al Presidente di recuperare il tempo che la volgarità e la maleducazione di Gasparri mi ha sottratto. Il tempo lo recupera il senatore Renzi, non vi preoccupate. RENZI *(IV-C-RE)*. Ho da dire una cosa al Partito Democratico: noi ieri abbiamo votato insieme. Se tutto il campo largo avesse votato insieme, la sinistra radicale, il MoVimento 5 Stelle, voi e il nostro Gruppo, noi avremmo avuto oggi un dato di fatto oggettivo: il Governo sarebbe andato a casa. casa. Nessuno ha il coraggio di fare i conti, perché mentre la Presidente del Consiglio può dire mi rimetto al voto del Parlamento, se il pensiero espresso dal Governo va sotto in Aula, il Governo va a casa. Allora, è legittimo salvare il Governo, è legittimo, collega Patuanelli, fare la stampella al Governo; quello che non è legittimo, amici del Partito Democratico, è non chiarirvi su questo punto, perché prima o poi anche per voi verrà il *redde rationem*. Volete stare con uno schieramento europeista coerente con quello che dice il vostro Commissario europeo, onorevole Paolo Gentiloni, coerente con la linea riformista che i vostri Governi hanno sempre espresso o pensate di inseguire un populismo sovranista, che critica la maggioranza soltanto perché aveva due posizioni diverse sul MES? Il campo largo ne ha avute tre di posizioni diverse sul MES e da questo punto di vista o fate chiarezza al vostro interno, o non vincerete mai. conclusione, Presidente, c'è un punto banale che voglio sottolineare e che affido alla Presidenza del Senato: per il quinto anno consecutivo, la legge di bilancio viene votata da un solo ramo del Parlamento, o meglio in prima lettura soltanto da ora, ma poi non ci sono le correzioni. Io sono favorevole al superamento del bicameralismo; ci vuole una riforma costituzionale se continuiamo con la consuetudine che questo Parlamento ha superato il bicameralismo senza dirlo, stiamo facendo un pessimo servizio alla politica, perché la politica non è dire ai *social* quello che ai *social* piace. La politica è avere il coraggio di fare battaglie scomode e la riforma costituzionale è una di queste: non più rinviabile. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signori del Governo, di questa manovra di bilancio si parla dal mese di agosto. Ovviamente era stata venduta come una una legge di bilancio che doveva favorire la crescita, aiutare i fragili, aiutare le famiglie, accrescere la giustizia sociale e sostenere il tessuto produttivo. Questa era la ricetta di cui parlava la Presidente del Consiglio, quale diceva anche che questa manovra di bilancio non doveva avere emendamenti, perché bisognava approvarla in fretta, entro il 28 novembre al Senato ed entro il 15 dicembre alla Camera in doppia lettura.

un voto di fiducia: questo è il dato fondamentale. Altro che due letture in tempi rapidi; in più stiamo votando un maxiemendamento di 561 commi.

che non è in grado di dare risposte al Paese. Non serve una legge di bilancio che non favorisce la crescita, che non aiuta i fragili, che non investe sulle famiglie, accresce il accresce il divario sociale - questo è il dato - e non dà risposte al tessuto produttivo, perché queste sono le questioni. L'ho detto già ieri e lo recupero oggi: secondo voi, qual è la risposta che dà questa legge di bilancio sul terreno delle politiche industriali, sul futuro del nostro sistema imprenditoriale; all'Ilva, alla TIM, all'ex Alitalia e a centinaia di aziende in crisi?

superbonus ha utilizzato una legge dello Stato che doveva essere applicata e oggi molte imprese si trovano in difficoltà perché non si offre una soluzione.

altri problemi dal punto di vista occupazionale. Sul terreno sociale, avete utilizzato i soldi della coesione sociale per programmare un'opera inutile come quella del Ponte sullo Stretto:

«disuguaglianza» non esiste. Avete cancellato il reddito di cittadinanza e non c'è un sistema universale. Avete scaricato sulle comunità locali la responsabilità di dare risposta alla questione del disagio sociale. E questo obbligherà i Comuni ad aumentare le tasse per dare una risposta. Vi lavate la coscienza scaricando su altri la responsabilità.

Quindi, bisogna fornire i servizi, come ad esempio gli asili nido. In questa legge di bilancio c'è una sola voce su un asilo nido in uno sperduto paese.

Questo significa che non è vero che mettete tre miliardi in più, certo nominalmente sì, ma riducete di sette miliardi la spesa sanitaria; se voi arrivaste al 6,9 per cento, ci vorrebbero 143 miliardi, e non

minimo è un modo per alzare la capacità di spesa dell'insieme del Paese e quindi trasferire i soldi dal capitale al lavoro. Questo è il dato fondamentale. È vero, ministro Giorgetti, che utilizzate 14 miliardi per il cuneo fiscale. Per fortuna pensate al cuneo fiscale. Ma, per risolvere questo problema, avreste dovuto affrontare il dato

diceva il sottosegretario Freni - che sono contenti di aver fatto una legge di bilancio politicamente orientata. Ora, c'è una differenza - anch'io sono contento da questo punto di vista - perché la destra pensa "ognuno per sé e Dio per tutti",

è grave. Durante l'intervento del presidente Renzi si è sentita chiaramente - lo ha colto tutta l'Assemblea - una frase ingiuriosa del presidente Gasparri nei confronti del presidente Renzi. Le chiedo di intervenire ai sensi del nostro Regolamento e le domando se la Presidenza possa consentire che, durante l'intervento di un collega,

Fatti e non bugie su questa manovra di stabilità. Per quanto riguarda il lavoro, 10 miliardi per il taglio del cuneo fiscale, che vuol dire aumento del salario reale, ed è il secondo anno che avviene; un aumento di 100 euro medi a testa. La Banca d'Italia - cito una fonte autorevole - ha calcolato poi che, con gli interventi fiscali, la delega fiscale e l'avvio di altre riforme, il vantaggio medio per le famiglie è pari euro l'anno. Il lavoro - parto da questo - è un tema fondamentale, perché non c'è altra politica sociale che quella di creare lavoro. Qualcuno pensava di risolvere tutto con l'assistenzialismo del reddito di cittadinanza. Invece oggi, senza reddito di cittadinanza, con il sostegno ai veri deboli,

750.000 posti di lavoro (buona parte dei quali a tempo indeterminato), ed è un *record* di occupazione dal 2004 ad oggi; il tasso di disoccupazione sceso intorno al 7 per cento. Il Gruppo Forza Italia, con la cultura dell'impresa e la cultura del lavoro, crede che la politica sociale migliore sia questa: creare occupazione e far uscire dalla marginalità sociale chi non aveva un lavoro. i soldi per il contratto del pubblico impiego - c'è qui il ministro Zangrillo - sono pari a otto miliardi nei prossimi tre anni. Ciò vuol dire contratti: lavoro, lavoro, lavoro. Questa è la prima risposta *(Applausi)* che noi diamo alla pubblica opinione con la legge di stabilità e la politica complessiva del Governo. Abbiamo poi altri dati. Questo Governo non doveva fare la legge di stabilità l'anno scorso, quest'anno non lo doveva fare, facendola come l'anno scorso il 28 e 29 dicembre. L'anno ha 365 giorni, tutti sono buoni.

La no tax area è stata estesa fino a 8.500 euro. Si è intervenuti sui *fringe benefit*. Sono state attuate semplificazioni. Si è avviata la riforma fiscale. Sono stati previsti famiglie con figli e interventi a favore delle madri che hanno tre figli e quant'altro. Ricordo il coraggio, non con la legge di stabilità, ma con l'avvio della riforma fiscale, di introdurre in Italia la Global minimum tax per far pagare finalmente qualche tassa ai giganti della rete che non pagano nulla. *(Applausi)*. Paga l'artigiano, paga il commerciante e non pagano Amazon, Google e Facebook. Questo Governo sta anticipando l'Europa e ha il coraggio di affrontare

a stilare l'elenco dei residenti illegali nelle case popolari. *(Applausi)*. Fa lo sceriffo in televisione, ma non sa fare neanche l'amministratore di condominio e il Governo sta risanando quella periferia, come altre. Anche questo rientra nella politica economica. Per quanto riguarda la sicurezza abbiamo varato, oltre alle misure per i nuovi contratti, un emendamento apposito. Mentre altri volevano fare marchette qui e là, abbiamo destinato 113 milioni alla specificità del comparto sicurezza e difesa, alle pensioni dedicate a questo settore. *(Applausi)*. Abbiamo preferito il popolo in divisa a Casarini e alle ONG degli amici di altri Gruppi parlamentari. Anche questo lo rivendichiamo come Forza Italia.

votato la riforma del MES, perché non ci facciamo dettare le scelte da altri. Antonio Tajani, vice presidente del Consiglio e nostro segretario, un europeista tra i più noti, ha detto più volte che il MES così non va, perché c'è una mancanza di democrazia e perché serve un controllo da parte del Parlamento europeo. Per questo ci siamo astenuti e l'abbiamo detto fin da quando lo diceva Berlusconi. Quindi, caro Presidente, noi in quest'Aula, fatte le scuse a chi le deve avere, lezioni

quando ci fu l'ingiusta decadenza di Berlusconi: quando c'è una sentenza definitiva, la partita è finita. Lo disse un senatore presente in quest'Aula: *game over* nei confronti di Berlusconi. Potevano applaudire Berlusconi da vivo e non usare in maniera distorta le sue parole oggi che Berlusconi non c'è. *(Applausi)*. Presidente, cito atti parlamentari; l'espressione *game over* ce la ricordiamo. Dopodiché, se qualcuno fa calare i voti del suo partito più rapidamente di quanto cali l'inflazione, non è colpa nostra. *(Applausi)*. E parla solo degli altri, per non parlare di se stesso. Siccome mi sono scusato, posso dire quello che penso. penso. Di fronte a lezioncine di questa natura, il Parlamento è libero, ognuno può dire quello che vuole e anche noi possiamo rispondere. Sull'Europa - lo dico a tutti, anche ai colleghi della maggioranza - il MES così

riscritta e rivissuta, serve, cari colleghi. Pensate che la Lorena, la Catalogna o il Molise da soli possano reggere il confronto non dico solo con gli Stati Uniti o con i Paesi del petrolio, ma anche con l'India, che quest'anno ha superato come popolazione la Cina, o con la stessa Cina e con la sua concorrenza sleale? L'Europa serve, ma serve un'Europa che difenda gli europei e che non sia fatta solo di regole burocratiche. *(Applausi)*. Noi a questo crediamo, per difendere le regioni e i territori dell'Europa,

la fiducia al Governo, che se l'è guadagnata sul campo; la fiducia a questa manovra di bilancio e alla politica economica complessiva. Certamente ci sono altri argomenti che avrei potuto citare, ma penso che i temi del lavoro, del taglio delle tasse, dell'avvio della delega fiscale, del sostegno alle famiglie, degli interventi per la sicurezza, la vicenda dei contratti del pubblico impiego e tante altre portino anche la firma di Forza Italia, dei nostri esponenti di Governo e della nostra coalizione, che è unita. Su alcuni grandi temi si sono divisi tutti ieri nella discussione alla Camera, non è che il dibattito c'è solo nella maggioranza. Ho voluto citare Silvio Berlusconi, perché noi siamo i custodi di quell'insegnamento politico, caro Presidente. E riteniamo che Forza Italia, in questi mesi di assenza del nostro presidente Berlusconi, abbia dimostrato la vitalità, la necessità e la indispensabilità del nostro movimento politico, che alle elezioni europee

per portare avanti queste politiche, che hanno creato lavoro e stanno creando condizioni migliori per un'Italia che ha tanti problemi. Voteremo la fiducia e onoreremo noi la memoria di chi va ricordato. E, se ci sono delle riconversioni postume, le accoglieremo con cristiana e fraterna comprensione. Meglio sposare le buone cause in ritardo che perseverare nell'errore. *(Applausi)*. La ringrazio, Senatore Gasparri, anche per aver attenuato la polemica di prima.

Dovevate, secondo voi, insistere sul no al MES per ottenere buoni risultati sul Patto di stabilità, che era in revisione a livello europeo. Ma di questa vostra strategia oggi non rimane nulla: un Patto di stabilità talmente lacrime e sangue per l'Italia che perfino l'Olanda ha festeggiato. Nemmeno i giornali di destra sono riusciti a difendere la scelta del Governo di dare l'assenso alla riforma del Patto di stabilità. Vorrei poi calare un velo pietoso sulla conferenza stampa dei Ministri tedesco e francese, che il nostro Governo ha seguito in *streaming,* in cui hanno comunicato l'avvenuto accordo: hanno detto che il Governo italiano è stato informato. Ringraziamo l'Europa per questa concessione, ci hanno informato. Il nostro ministro Giorgetti ripeteva fino al giorno prima che il Patto, così come approvato oggi, non è adatto per un Paese ad alto debito come il nostro. Insomma, un disastro. Ci avete raccontato che l'Italia era tornata centrale, credibile a livello europeo. La verità è che questo Governo porta non soltanto all'isolamento del nostro Paese, ma ci obbliga anche a prendere schiaffi e a dire anche grazie a chi ce li sta dando. Siamo umiliati, schiaffeggiati e ricattati dall'Europa. Tornano vincoli rigidi, parametri contabili prociclici, una nuova stagione di austerità. Bisognava invece difendere la politica che ha consentito, in una fase di grande complessità economica per tutta l'Europa, di portare debito comune europeo e 200 miliardi al nostro Paese. Questo andava fatto: andava difesa la dignità del nostro Paese. Il tutto si conclude con il comunicato di Palazzo Chigi in cui si esprime rammarico per l'approvazione di un patto a cui abbiamo dato l'assenso. Io vorrei manifestare la massima solidarietà al ministro Giorgetti, perché penso che che suscitare rammarico nel Governo di cui si fa parte sia sicuramente poco piacevole. Per uscire da questo *tunnel* in cui avete infilato il Paese per i prossimi decenni, però, il colpo di scena finale è stato il voto MES. Non vi siete accorti, tuttavia, che le condizionalità del MES, le automazioni di quel meccanismo, il rientro automatico del debito e la compressione del *deficit*, le infrazioni e le multe per i Paesi ad alto debito sono di fatto entrate a spron battuto nel Patto che è stato approvato con le modifiche al Patto di stabilità. Ci ritroviamo con un Patto di stabilità lacrime e sangue e con il vecchio MES ancora in piedi, quello del 2011, quello che avete fatto voi. Oggi è calata la maschera: tutti i parametri europei, dal MES del 2011 al nuovo Patto di stabilità, sono figli di un Governo di destra, che porterà danni enormi a questo Paese. Più che sovranisti, siete sovranisti a sovranità limitata. *(Applausi)*. Passando alla manovra, citerò in questa parte di intervento una frase che è divenuta un mantra del Presidente del Consiglio. Recentemente in quest'Aula ha detto che c'è la propaganda poi ci sono i documenti. L'ha detto sventagliando un fax che evidentemente non aveva letto, ma questa è un'altra storia. Dati alla mano e considerando anche il crollo delle economie europee del 2020, la crescita del PIL

perché c'è la propaganda e poi ci sono i documenti. Continuando con i dati, D'altronde, siete il Governo dello zero virgola. Ma questo significa che l'unico vero buco di bilancio per il 2024 non è il superbonus, ma è quello che fate voi con il Documento di economia e finanza e una previsione di bilancio che parla di crescita all'1,2 per cento quando la crescita reale sarà dello 0,6

dice che non butta via i soldi degli italiani dalla finestra. Va bene, ma i soldi li va a prendere direttamente dalle tasche degli italiani. Citiamo alcuni dati: 21 miliardi di tagli alle pensioni dei dipendenti pubblici; 37 miliardi di tagli in diciassette anni all'indicizzazione delle pensioni; aumento delle tasse su pannolini, assorbenti, latte in polvere; cancellazione delle agevolazioni fiscali; cancellazione degli sgravi per gli *under* 36 che acquistano la prima casa; umiliazione del piano Transizione 4.0 (altro che industria); cancellazione della detrazione IVA al 50 per cento per chi acquista case con classi energetiche superiori; tagli alla sanità; tagli all'istruzione; cancellazione dello sconto in fattura tranne per i bagni e, quindi, avete introdotto il superbonus del water. Sul superbonus, dico soltanto due cose, perché non voglio riaprire La presidente Meloni ha detto che qualcuno prima o poi dovrà fare i conti con la propria coscienza per aver immaginato così male un provvedimento, tanto da trasformarlo nel più grande regalo mai fatto dallo Stato italiano a truffatori e organizzazioni criminali. i decreti attuativi del superbonus hanno la mia firma: nessuno può permettersi di dire a me e alla mia forza politica di aver fatto una misura per aiutare criminali e truffatori di questo Paese. Nessuno può permettersi di dire una cosa del genere.

che, se non si fanno investimenti per le imprese, la crescita non c'è; nove mesi consecutivi di calo della produzione industriale in termini tendenziali; investimenti crollati, +20 per cento nel 2021, 10 per cento nel 2022, 0,6 previsto nel 2023 e nel 2024 perché c'è la propaganda e poi ci sono i documenti. Sul cuneo fiscale, è una mera riproposizione di qualcosa che c'è, giusta, sacrosanta, ma non si possono illudere gli italiani che da gennaio avranno 100 euro medi in busta paga in più e 600 euro medi nell'anno, perché la busta paga di gennaio sarà identica a quella di dicembre. *(Applausi)*.Quell'aumento è totalmente mangiato dall'inflazione, perché c'è la propaganda, ma poi ci sono i dati. Avete imposto al Paese la litania della coperta corta, con la destra l'Italia è sempre l'ultima della classe, quella a cui mancano i soldi per fare qualsiasi cosa. Non cito per decenza la storia della tassa sugli extraprofitti, perché è una figuraccia che si commenta da sola. La realtà che sta emergendo è che avete il terrore negli occhi, perché l'ultimo Governo italiano di centrodestra ha portato lo *spread* a 5,75, le conseguenti dimissioni del Presidente del Consiglio per evitare il *default*, e questo vi sta togliendo il coraggio. Eppure noi, quelli del buco di bilancio, dell'incapacità, dell'incompetenza abbiamo affrontato la più grave crisi economica della storia di questo Paese, portando un'economia più solida di come l'abbiamo trovata e contemporaneamente avevamo uno *spread* sotto i 100 punti base. Evidentemente, le agenzie di *rating*, i mercati, le borse, lo *spread* non si erano accorti del danno che avevamo prodotto durante la pandemia e ci hanno pure dato in Europa più di 200 miliardi. Pensate un po'. Come ho detto tutto il tempo, c'è la propaganda e poi ci sono i documenti. La differenza è che i nostri documenti sono veri, mentre quelli che sventolate voi in quest'Aula sono documenti falsi. Ovviamente, la colpa di tutto questo non è vostra, la colpa è dei benzinai, della Wagner, della Lagarde, delle crisi geopolitiche, della magistratura, e ovviamente del superbonus, perché avete trovato la scusa per i tagli che dovrete fare per i prossimi quattro anni. Peccato che oggi - sempre per citare i dati - è arrivata la prima stima di cosa significheranno i tagli del pacco di instabilità e decrescita che avete votato. L'istituto Bruegel parla di una correzione minima di 12 miliardi l'anno se le cose vanno bene e dal 2027 sarà ancora peggio. Significa un miliardo di euro al mese di tagli, 48 nel corso della legislatura. E con la crescita prossima allo zero, senza la possibilità di usare il *deficit*, la domanda è dove troverete un miliardo al mese di tagli se non tagliando i servizi che lo Stato garantisce agli italiani. Avete detto che non avreste mai dato l'ok a un accordo impossibile da rispettare. L'avete fatto e vi faccio i miei migliori auguri per questo. A proposito di auguri, siamo in un clima natalizio, è il momento in cui si sognano i regali da mettere sotto l'albero. Per me, per noi, per il mio Gruppo, per l'opposizione di questo Paese, per i cittadini e per il Paese chiedo soltanto un regalo: che ve ne andiate il prima possibile.

una grossa caduta di tono che mi sento di censurare. internazionale particolare, coda di pandemia, inflazione, guerre, incertezza sui mercati, il dato politico di questa manovra si riassume in due punti. Il primo è rappresentato dal fatto che usiamo le poche risorse a disposizione che abbiamo non per creare nuova spesa, ma per ridurre le tasse ai più bisognosi. Questo è il primo tema che mettiamo in risalto. *(Applausi)*. In secondo luogo, abbiamo di fronte una manovra fatta con responsabilità, serietà, prudenza, che ci ha fatto superare l'esame dei mercati, ponendo l'Italia in un contesto di credibilità internazionale, a dispetto di coloro che pensavano che questo Governo sarebbe durato solo sei mesi. nonostante le difficoltà che abbiamo incontrato. Indubbiamente, i crediti d'imposta da superbonus e il rialzo dei tassi hanno fatto mancare alle casse dello Stato circa 35 miliardi di euro. Questi avrebbero potuto, sì, essere utilizzati per tante altre misure, ma non abbiamo potuto farlo. È una manovra di bilancio bilancio con un aspetto molto sociale, orientata ai ceti medio bassi, prevalentemente ai lavoratori dipendenti. Certo, la conferma del taglio del cuneo fiscale è un'ottima misura. L'anno scorso io sentivo, da parte delle opposizioni - ai tempi erano nel Governo Draghi - interventi di giubilo per i due punti di taglio che il Governo Draghi aveva fatto senza neanche metterli a livello strutturale. Oggi, però, che questo Governo di centrodestra conferma il taglio fino a sette punti, allora no, non va bene, bisognava renderlo strutturale. Diciamocelo chiaramente: non va bene perché non l'avete fatto voi e l'ha fatto un Governo di centrodestra. Ma possiamo parlare anche della riduzione dell'aliquota Irpef dal 25 al 23 per cento per i redditi che vanno da 15.000 a 28.000 che sarà anche propaganda, ma è stata Banca d'Italia a dire che, in media, ci saranno 600 euro in più in busta paga per tre famiglie su quattro. Se l'ha detto Banca d'Italia, sarà anche propaganda, ma probabilmente qualcosa di vero c'è.

della *no tax area*, sempre per i dipendenti; ai sette miliardi che mettiamo sul rinnovo dei dipendenti della pubblica amministrazione. Anche questo è un segnale importante e decisivo. Ancora, cito la rivalutazione delle pensioni al 5,4 per cento, fino a quattro volte le minime. comprendiamo dall'opposizione un po' di prurito, perché mai un Governo di centrosinistra aveva fatto una manovra così attenta nei confronti dei ceti medio bassi come sostanzialmente abbiamo fatto noi. Compagni, su col morale, in fondo stiamo realizzando i vostri sogni. *(Applausi)*. Certo, non tutto va bene. Ci sono stati anche degli incidenti di percorso, come sicuramente la questione delle pensioni dei medici, su cui poi il Governo è intervenuto, sostanzialmente per scongiurare i tagli inizialmente previsti per medici, dipendenti degli enti locali, ufficiali giudiziari ed altre Certo, sulla sanità avete ragione quando dite che il fondo andrebbe valutato al netto dell'inflazione. Ma non era scontato che questo Governo, con le difficoltà che ha incontrato, mettesse tre miliardi sulla sanità e prevedesse degli interventi a progetto per ridurre le code sulle liste d'attesa. Qualcuno ci ha detto che abbiamo fatto poco per le imprese. Qualche misura interessante di sicuro c'è: la superdeduzione fino al

chi conosce bene i territori sa quanto siano importanti. E cito poi due misure che ha voluto fortemente la Lega, che sono le nuove regole sul Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese,

che ha trovato, insieme al ministro Giorgetti (un Ministro e un Sottosegretario della Lega), le risorse necessarie per dare ancora spazio alle nostre piccole e medie imprese. fatto - a cui teniamo particolarmente - che finalmente siamo riusciti a spostare l'acconto fiscale di novembre al nuovo anno, con un pagamento in un'unica soluzione a gennaio, o la possibilità di rateizzare fino a giugno, dando un segnale importante anche a professionisti e partite IVA. Certo, qualcuno ci ha detto che abbiamo fatto poco per la crescita. Ho sentito in qualche vostro intervento dire che vi aspettavate un po' più di coraggio, che manca una visione in questa manovra e che questa è una legge di bilancio costruita sul solco dell'ideologia dell'austerità. A parte che mi meraviglia un po' che arrivino questi strali e queste critiche sulla troppa austerità della manovra da parte di chi dell'austerità in Europa per anni ha fatto una propria bandiera. Poi, se mi permettete, oggi avere coraggio significa principalmente sistemare i conti dello Stato. Avere una visione significa non lasciare dei buchi di bilancio per quelli che verranno dopo. Questo è un modo diverso di guardare le cose con attenzione, a differenza di come succede di solito: si spendono le risorse avvelenando i pozzi per quelli che verranno dopo. Che cosa volevate? Volevate un aumento sconsiderato della spesa corrente, come ha chiesto anche qualche sindacato? Vedete, una politica più espansiva indubbiamente avrebbe esposto il nostro Paese a una

che sono stati toccati in chiusura di dichiarazione di voto: uno è la questione degli extraprofitti sulle banche, su cui qualcuno dice che è stata fatta una figuraccia. In realtà, noi pensiamo che non si sia trattato assolutamente di una retromarcia, al di là di quelle che possono essere state considerate alcune dichiarazioni roboanti iniziali.

terra quelli che sono i desideri e i sogni di qualcuno che, sì, la propaganda probabilmente la sta facendo. Ma noi siamo corretti fino in fondo, perché anche sul superbonus, al di là del fatto che è stata la misura di bandiera di bandiera del MoVimento 5 Stelle, sarebbe il caso di dire in quest'Aula, visto che abbiamo seguito tutte le numerose manovre: chi non ha peccato scagli la prima pietra. Forse una pietra potrebbe tirarla il ministro Giorgetti, che dall'inizio di questa vicenda ha sempre riconosciuto con estrema chiarezza che c'era un grosso problema su questa misura. La prossima volta un po' tutti dovremmo stare decisamente più attenti. Naturalmente un pensiero non può che venire, in fase di chiusura,

alla sovranità che appartiene al Parlamento italiano. *(Applausi)*. Di questo bisognerebbe essere felici, anziché arrabbiarsi, come ha fatto qualcuno di sinistra, che ha un concetto di democrazia un po' strano: se il voto va nella direzione gradita, allora la democrazia è stata rispettata; altrimenti, non va assolutamente bene.

Mi fa piacere salutare insegnanti e studenti dell'Istituto comprensivo «Giacomo Matteotti» di Riano, vicino Roma.

Signor Presidente, la seconda legge di bilancio del Governo Meloni impone, colleghi della maggioranza, signori del Governo, ancora più nettezza di quella che questo Parlamento richiede in momenti cruciali: sono passaggi in cui il Paese si guarda allo specchio e prova a capire se la politica riesce a dare risposte a istanze molto complesse.

presente con lo spirito in tutte le nottate e le giornate di lavoro della Commissione bilancio. Signor Presidente, questa manovra ci preoccupa perché è scritta sull'acqua. perché è scritta sull'acqua. Colleghi, per la seconda volta consecutiva in due anni scrivete una manovra basata su previsioni errate. Nel 2022 avevate previsto una crescita del Paese che poi avete completamente corretto. Non paghi di tutto questo, vi siete presentati in Parlamento signor Ministro, deve spiegarci come farete - dicendo che cresceremo dell'1,2 per cento. Il PIL programmatico, solo per il Governo Meloni, è dell'1,2 per cento.

La nostra preoccupazione è tutta legata a quello che avete messo dentro la manovra, perché è improntata sul breve termine in un contesto fragile e incerto, con poche risorse a disposizione. Al presidente Romeo, che ha ricordato mirabolanti interventi, dicendo che non c'erano risorse e che non potevano far altro, vorrei ricordare che avete scelto di non prendere risorse, perché di lotta all'evasione infatti non c'è nulla *(Applausi)*: avete infatti ribadito il solito approccio della destra sui condoni e avete proposto rottamazioni non per gli italiani o e le italiane in difficoltà,

su cinque che ha questo impianto non poteva certamente essere costruita su due pilastri che hanno un inizio e una fine con l'anno 2024. È questo quello che ci preoccupa di più, perché sono nettamente aumentati i rischi al ribasso per l'anno prossimo, la produzione è in frenata, il nostro PIL non si espande da un anno, c'è un'evidente deterioramento della domanda interna e i consumi delle famiglie hanno esaurito la fase di recupero successivo alla pandemia: e voi cosa fate? Mettete 11 miliardi su una misura che vi avevamo chiesto di rendere strutturale, il cuneo fiscale, sapendo che l'anno prossimo si partirà non solo da -11 ma da -15. Da quest'anno, chiunque si sieda sulla scrivania del Ministro dell'economia - non sappiamo quanto resterà dopo i silenzi legati alla riforma del Patto di stabilità e alla mancata ratifica del MES - per fare una manovra nel nostro Paese, partirà da -15. Siamo tornati alle clausole di salvaguardia del 2008-2011. Siete sempre gli stessi. Molti dei Ministri di questo Governo c'erano anche allora. Allora in ostaggio c'erano i consumatori (ricordate gli aumenti dell'IVA nel caso in cui non accadessero alcune cose?), ora in ostaggio ci sono i lavoratori, ora in ostaggio ci sono gli italiani e questo non ve lo potevamo consentire, perciò l'abbiamo contestato. Per questo abbiamo detto più volte: fermatevi e lavoriamo insieme per rendere quelle misure strutturali. Non si è mai vista in Italia, ministro Giorgetti, una riforma fiscale che accorpa due aliquote ed è a tempo determinato: un anno. Cosa succederà l'anno prossimo? *(Applausi)*. Cosa diciamo a chi oggi pagherà il 23 per cento per l'anno prossimo? Non lo sappiamo: dipenderà dalla congiuntura, da quello che accadrà e da quello che succederà. È scritta sull'acqua, ma non è l'acqua di Neruda, perché ad un certo punto, nelle tante giornate passate insieme in Commissione bilancio, abbiamo pensato che, come Neruda, vi faceste tante domande andando a vivere sulla riva del mare. Lui gettava quelle domande in acqua, perché le risposte avrebbero fatto litigare tutti. Voi avete deciso di dire al Paese che, siccome non c'era altro da fare, siete diventati all'improvviso austeri. No,

È un gravissimo passaggio graduale dalle pensioni di anzianità a quelle di vecchiaia. *(Applausi)*. Avete approfittato della condizione di debolezza di centinaia di migliaia di italiani e gli avete detto: decidiamo noi. Poi avete scoperto che c'erano i medici tra quei 730.000 italiani, e siccome c'erano i medici avete fatto marcia indietro. È venuta qui la Presidente del Consiglio ad ammettere che era uno sbaglio, ma la toppa è stata peggiore del buco, la toppa è stata peggiore del buco, soprattutto quando avete dovuto prendere atto dell'umiliazione che avevate inflitto al Parlamento invitando a non presentare emendamenti, dovuto finire il 15 dicembre. Siamo al 22 dicembre, non abbiamo ancora fatto il primo voto qui al Senato. Ve lo dico e lo sottolineiamo, perché quando vi abbiamo chiesto, sperando che in qualche modo ci fossero un moto o un sussulto di dignità,

Abbiamo assunto un impegno per dare un segnale al Paese. Sappiamo benissimo che non bastano 40 milioni per fermare il dramma della violenza di genere, ma era un segnale e speravamo di poterlo fare insieme. Avete perso anche questa occasione. non è quella che raccontate. L'Italia, signor Presidente, non meritava le umiliazioni a cui noi abbiamo fatto fatto riferimento nel dibattito che abbiamo svolto in Aula. L'Italia non è quella che raccontate nell'accordo capestro fatto con l'Albania. Questi sono i numeri dei migranti, signor Presidente; siamo passati da 64.000 a 153.000 e non è cambiato nulla, la condizione di questi quattordici mesi è peggiorata. abbiamo contestato in queste ore la postura del nostro Paese in Europa non solo perché il nuovo Meccanismo europeo di stabilità, che l'Italia non ha ratificato, nasceva dal fondo del del vecchio salva Stati e quella riforma dolorosa che aveva portato al salvataggio della Grecia era stata abbondantemente superata. Lo abbiamo fatto perché abbiamo seguito con attenzione la dinamica che aveva portato lo stesso ministro Giorgetti ad essere silente in Europa durante la trattativa della riforma del Patto di stabilità. Ministro Giorgetti, l'Italia era stimata e rispettata in Europa e lei lo sa, perché è stato in ben due Governi su tre dell'ultima legislatura. Oggi è l'Italia del fingere di fare per non fare nulla, è l'Italia inaffidabile contro cui si sono battuti gli italiani,

della maggioranza sovranista, non può essere considerato un ostacolo alle politiche nazionalistiche o un intralcio a disegni propagandistici contro ogni forma di integrazione. l'Europa è stata un'idea straordinaria di comunità, una grande idea di pace, di moderna prosperità, per un mondo in continua evoluzione, grazie al progresso.

signor Presidente, l'Europa non è un incidente della storia, come ci ricordava David Sassoli, che dovreste sempre e comunque avere come stella polare.

Proprio David Sassoli ci ha insegnato che questa è la nostra più grande speranza: non vi consentiremo di tradirla e vi metteremo di fronte alle vostre responsabilità. *(Applausi)*. PRESIDENTE.

per noi sono molto importanti. Come dicevo, questa è una legge di bilancio coraggiosa, che noi di Fratelli d'Italia e di tutto il centrodestra abbiamo apprezzato, perché abbiamo avuto la forza, il coraggio e la serietà, in un momento delicato e difficile per il Paese, di approvare una legge di bilancio che guarda all'interesse della Nazione e non si limita

da chi prima di noi ha dilapidato decine e decine di miliardi per misure elettoralistiche *(Applausi)*, che hanno fatto male al nostro Paese e hanno messo in disequilibrio i conti dello Stato e i conti del MEF. Questo è il grande problema su cui oggi dobbiamo ragionare. Come dicevo, questa legge si presenta in un momento da tempesta perfetta. Non

ma abbiamo subito anche di peggio dal punto di vista economico, con l'Italia bloccata per lunghissimi mesi, per più di due anni, con tutto il suo apparato produttivo.

conflitti hanno messo in evidenza un problema importante di crisi energetica, che ha dimostrato tutti i limiti dei Paesi europei negli scorsi decenni e su cui il Governo Meloni da un anno e due mesi sta cercando di recuperare, per dare una prospettiva nuova al nostro Paese. Ricordiamoci però anche cos'è accaduto con la scorsa legge di bilancio. Signor

20 dei quali sono stati impegnati per le famiglie e le imprese italiane, per il caro energia e per il caro bollette, per sostenere il sistema economico e sociale del Paese. Queste sono cose che purtroppo si dimenticano molto spesso. L'indicazione è stata chiara lo scorso anno, quando abbiamo fatto scelte precise; e siamo stati ancora più chiari quest'anno, quando abbiamo fatto quadrato intorno ai nostri connazionali e abbiamo aiutato le persone che oggi soffrono. Aiutiamo gli ultimi e tutti colori che hanno difficoltà, perché in questo momento tutto il resto passa in secondo piano. Ci sono pilastri su cui abbiamo lavorato.

Le chiedo quale sia lo scandalo, se una maggioranza che si riconosce in un Governo politico decide di supportare l'azione della propria maggioranza. Cosa c'è di tanto scandaloso, senatore Renzi? Noi siamo stati d'accordo nel sostenere il progetto di bilancio presentato dal Governo Meloni, che segue una direzione chiara quanto ai pilastri del lavoro, delle pensioni, delle famiglie e delle imprese.

non sono le indicazioni che diceva il collega Renzi rispetto ai 18 miliardi del patto di stabilità, ma derivano dai 20 miliardi di superbonus che pesano fortemente sulle casse dello Stato

europea. Nella formazione di questa manovra di bilancio siamo quindi partiti da -35 miliardi di euro; nonostante tutto questo, però, le risorse le abbiamo trovate, anche se in parte sono in *deficit*, dando priorità, come ho già detto, agli italiani che in questo momento stanno facendo più fatica ad andare avanti.

fiscale e contributivo dei dipendenti pubblici e privati italiani, una platea di 14 milioni di contribuenti, che vale 10 miliardi di euro.

Sul lavoro abbiamo detassato i *fringe benefit* fino a 2.000 euro per chi ha figli a carico; abbiamo ridotto la tassazione per i premi di risultato dei dipendenti delle aziende private e interveniamo ancora sulle pensioni;

Giorgetti. Dovevamo sovrapporre il Piano nazionale di ripresa e resilienza al bilancio che ci stiamo apprestando ad approvare, perché quella montagna di risorse sarà importante per dare uno sviluppo

che comincia a prendere forma, e l'attuazione di questo programma politico e del Governo è l'espressione di una visione chiara che abbiamo come Paese. la legge di bilancio 2024 fornisce i mezzi e gli strumenti per iniziare ad operare e a proiettarsi in un futuro, con l'auspicio di prosperità che

onorevole Giorgia Meloni mi ha mandato una breve lettera in cui scrive: «Nell'approssimarsi del santo Natale e dell'arrivo del nuovo anno, ti scrivo per esprimere tuo tramite a tutti i senatori e al personale in servizio presso il Senato della Repubblica i miei personali auguri e quelli del Governo». La ringrazio e ricambio. l'apprezzamento sul concerto di Natale, ma quello non ho bisogno di leggervelo. A questo punto, anche se ancora abbiamo un paio d'ore di lavoro, unisco miei auguri a tutti i senatori, ringraziandoli per l'impegno con cui, nella diversità delle posizioni, hanno trascorso questo anno politico. Come Come Presidente, non posso che rivolgere a voi, alle vostre famiglie e ai vostri affetti i migliori auguri di un Santo Natale e di un felice anno nuovo. presentato dal Governo, interamente sostitutivo degli articoli della prima sezione del disegno di legge n. 926, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.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

I senatori favorevoli alla fiducia risponderanno sì; i senatori contrari risponderanno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza. Estraggo ora a sorte

Invito il senatore Segretario a procedere all'appello, iniziando dal senatore Mazzella.

Proclamo il risultato della votazione nominale con appello dell'emendamento 1.9000, presentato dal Governo, interamente sostitutivo degli articoli della prima sezione del disegno di legge n. 926, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia:

poiché sono stati esaminati tutti gli articoli al disegno di legge, il Governo dovrà ora procedere alla stesura della conseguente Nota di variazioni, che sarà trasmessa al Senato non appena possibile. La 5a Commissione permanente è sin d'ora autorizzata a convocarsi per l'esame di tale documento e quindi a riferire all'Assemblea. In attesa della presentazione da parte del Governo della Nota di variazioni al bilancio, sospendo la seduta.

con la quale il Governo ha provveduto ad introdurre nel testo del disegno di legge e nelle annesse tabelle le modificazioni conseguenti alle determinazioni adottate dal Senato in sede di esame della prima sezione.

pochissimi attimi per il ricordo di una persona che è mancata questa mattina, Giancarlo Tesini. Bolognese, è stato a lungo parlamentare e a lungo Ministro della ricerca scientifica e dell'università, Ministro dei trasporti, consigliere comunale nella mia città fino agli anni '50. È stato un grande sportivo, presidente della Fortitudo e presidente della Lega Basket. È un uomo che ha lasciato un ricordo indelebile a Bologna, tra tutti coloro che l'hanno conosciuto e anche nella politica nazionale. Voglio ringraziare tutte le parti politiche, dal sindaco di Bologna ai principali esponenti dell'opposizione bolognese - sono ovviamente di Governo e della maggioranza nazionale - per i ricordi commossi che hanno avuto nei suoi confronti. Se lo meritava: è stato un uomo buono, onesto, giusto,

onorevoli senatori, la presente Nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026 è stata predisposta al fine di recepire nel disegno di legge di bilancio gli effetti degli emendamenti approvati dal Senato della Repubblica. In relazione a quanto precede, la presente Nota aggiorna i valori contabili dell'ex articolo 106 *(Totale generale della spesa)* del disegno di legge di bilancio e comporta modifiche: ai quadri generali riassuntivi per il triennio 2024-2026 in termini di competenza e di cassa; *b)* allo stato di previsione dell'entrata (Tabella n. 1) e a tutti gli stati di previsione della spesa dei Ministeri (tabelle da 2 a 16). Si producono in conseguenza anche le modifiche ai relativi allegati tecnici per capitoli. I prospetti sono organizzati per unità di voto e gli allegati tecnici per capitoli presentano l'intero bilancio dello Stato e con evidenza dell'unità e dei capitoli che hanno subito variazioni per effetto degli emendamenti al disegno di legge. Le variazioni connesse agli emendamenti approvati sono esposte in apposite colonne, distintamente per la Sezione 1 e la Sezione 2. La 5a Commissione ha conferito il mandato ai relatori a riferire favorevolmente all'Assemblea.

si intenderà modificato di conseguenza il testo su cui il Senato si è pronunciato nelle precedenti fasi della procedura, in riferimento sia agli articoli del disegno di legge, sia alle annesse tabelle.